Signor Presidente, onorevoli senatori, prima di tutto vorrei inquadrare questo decreto, questo complesso di norme,

Autorità e delle professioni, di norme sull'azione collettiva dei consumatori, sui servizi pubblici locali, sull'energia e così via.

delle nostre iniziative legislative o di questo stesso decreto, stiamo cercando di lanciare un messaggio riformatore un po' più ampio. Questo stesso provvedimento non si può leggere solo in chiave di liberalizzazioni in senso classico. Abbiamo in testa un'idea, che è un po' la c'è un collegamento fra economia e società, fra economia e diritti di cittadinanza, fra ruolo e dignità del cittadino consumatore; se la prendiamo dal lato del cittadino consumatore, diamo una mano anche all'ammodernamento e alla qualificazione dei nostri soggetti economici. economici. Per noi il punto di riferimento è che il cittadino non è un suddito e non può essere trattato come un suddito neanche da chi vende prodotti. Un giovane che vuole iniziare un'attività deve chiedersi se sa svolgerla e non chi conosce per poterla Le tasse bisogna pagarle per poterne pagare meno e per far questo non c'è bisogno tanto di carabinieri o finanzieri, ma di meccanismi, di una nuova fisiologia, come, ad esempio, la moneta immateriale. Chi fa impresa deve essere aiutato, non ostacolato, e così via. Ora, questi princìpi sono una sfida anche per noi, perché non è semplice essere coerenti con essi, però, però, l'insieme delle nostre norme ha questa ambizione, quella cioè di muovere le cose su una linea di riforma sulla quale ci piacerebbe poter avere un confronto culturale e politico di reciproca

Paese. Forse saranno stati anche limiti nostri, ma sull'insieme di queste attitudini non si è riusciti ancora a costruire una discussione, un dibattito politico, anche con le forze dell'opposizione, che ci portasse su un terreno di reciproca sfida.

proposito dell'umorismo che si è fatto sull'articolo che riguarda quella dozzina di professioni per le quali eliminiamo il vincolo di distanza minima, i numeri chiusi e così via. Sono, invece, norme che hanno avuto nell'opinione pubblica un rilievo significativo. Non so, infatti, chi si sentirebbe di andare a dire a un giovane, che ha speso 2.000 o

poca cosa. Solo in Italia si pensa che sia cosa piccola, perché, nella nostra implicita apologetica del corporativismo, ci siamo abituati a pensare: una corporazione cosa sarà mai? Non fa certo macroeconomia. E invece gli anglosassoni sanno che fa macroeconomia. Se andate a leggere la ricerca fatta dall'*Antitrust* sulla diversa applicazione della riforma del commercio in varie Regioni italiane, vedrete che l'effetto nella differenza della formazione dei prezzi è abbastanza impressionante.

Di più: noi non stiamo intervenendo sui prezzi e sulle tariffe; stiamo sostenendo, come nel caso della ricarica (ma vale lo stesso per il massimo scoperto) che si deve pagare quel che si consuma. In secondo luogo, non si può essere prigionieri di un servizio oltre il tempo tecnico e la spesa necessaria ad uscirne, se si intende uscirne. Questo è il principio. Si è detto che ciò poteva ben essere ovviato dal mercato, che non c'era bisogno di una norma. Condivido: poteva essere ovviato dal mercato. Se, per esempio, una compagnia telefonica, due anni fa, avesse avanzato una proposta

Ancora: si potrebbe obiettare che, se i famosi attori stranieri ed europei, che giustamente invochiamo quasi come una presenza che possa modernizzare il nostro assetto di concorrenza, portassero gli istituti che conoscono a casa loro, non vi sarebbe stato bisogno di queste norme. Invece, tutti si acquartierano, si mettono al calduccio, si rimpannucciano sotto le comodità che noi ancora forniamo.

Non facciamo il bene di queste aziende. Io credo che sollecitare delle novità sia il modo di tener in tiro un'economia che deve modernizzarsi, perché se le cose non sono così in Europa su una certa pratica, prima o poi non saranno così neanche da noi.

ma sono abbastanza stupito che ci sia stata una tale coralità, perché almeno l'anomalia di realizzare la più grande opera pubblica d'Europa senza una gara, neanche dall'inizio,

all'avvio di impresa con autocertificazione garantita da società professionali assicurate.

Allora, anziché venirsi a lamentare perché eliminiamo la tariffa minima, vediamo cos'altro possiamo fare in termini di modernizzazione delle professioni, visto che c'è un bisogno enorme di terziario professionale.

Il Governo, le Autorità, ma anche il Parlamento devono riuscire a guardare in modo unitario a questo tipo di problemi, forse anche sottraendoli

le misure, a nostro giudizio importanti per i cittadini, per introdurre ulteriori elementi di competitività che superino corporativismi nella società. Conoscete l'importanza che il Governo attribuisce a queste misure

alla Camera i Capigruppo dell'Unione - i Capigruppo di maggioranza - per due settimane hanno chiesto al Governo e al Ministro responsabile di porre la questione di fiducia, dicendo che non cera possibilità di confronto né di dialogo vero.

e tuttavia non possiamo far decadere queste misure. Vi sono due disegni di legge sulle liberalizzazioni: uno è stato

siamo alla quarta, con i disegni di legge, da parte di questo Governo. Quindi, vedremo se su tali temi questo confronto avrà luogo. Certo, non avrei mai immaginato - e questo è stato anche il mio errore - che

la scelta del Governo di porre la questione di fiducia. Queste sono considerazioni ed approfondimenti che dovremo svolgere e che io sento il bisogno di fare circa il rapporto tra le responsabilità del Governo e quelle del Parlamento. Oggi, però

non è ordinario. Allora, per tali motivi, a nome del Governo, autorizzato a questo dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1427, di conversione del decreto-legge, n. 7, del 2007, nel testo identico a quello approvato dalla Camera

all'organizzazione del dibattito sulla fiducia posta dal Governo sul decreto-legge in materia di liberalizzazioni. La discussione, per la quale sono state ripartite tra i Gruppi quattro ore, avrà inizio immediatamente,

In ogni caso, a partire delle ore 10 si passerà alle dichiarazioni di voto e successivamente alla chiama, che si presume avrà luogo intorno alle ore 11,45. Per quanto riguarda il decreto-legge sulla prevenzione della violenza nelle competizione calcistiche, la discussione già prevista per il pomeriggio di martedì 3 aprile, è anticipata allo stesso giorno alle ore 11. Gli ordini del giorno al bilancio interno del Senato - la cui discussione è prevista per la seduta antimeridiana di mercoledì 4 aprile - dovranno essere presentati entro le ore 12 di martedì 3 aprile. In apertura della stessa seduta, si svolgerà la chiama per la votazione relativa all'elezione di quattro componenti effettivi e di quattro supplenti della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, con il sistema delle urne aperte. È differito alla settimana dopo Pasqua l'esame delle mozioni sulla politica agroalimentare e sulla medicina di genere. Per il resto, il calendario corrente resta invariato.

pare per gentile concessione del Presidente della Commissione bilancio; peraltro, mi è stato detto dal funzionario che la relazione è ancora in bozza.

Al momento non sono pronti e questo mi sembra assolutamente inusuale

Il punto della nostra critica è che in quest'occasione si ripete lo schema del passato decreto Bersani-Visco. Anche allora, infatti, si trattò di lanciare in orbita le liberalizzazioni riguardanti le licenze dei taxi, la questione dei farmaci da banco e del ridimensionamento dell'attività dei notai. Eppure, subito dopo c'erano le terribili norme dovute alla fantasia di Visco per ridurre lo spazio di libertà nei confronti di tutti i cittadini

ministro del tesoro il presidente Ciampi, che stimo e a cui sono legato da sentimenti di sincera riconoscenza e apprezzamento, riguardò l'assegnazione delle licenze per la telefonia al gruppo Olivetti per 700 miliardi di L'Olivetti conferì queste licenze in una *joint venture* con la tedesca Mannesmann che prese la forma di una società olandese. Dopo circa un anno e mezzo, l'Olivetti vendette tale partecipazione al prezzo di 3.000 euro sempre alla tedesca Dopo alcuni mesi, la società Mannesmann fece acquistare queste quote alla Vodafone inglese che le incorporò. Così la Vodafone si trovò La licenza fissa per Infostrada fu successivamente rivenduta all'ENEL di Tatò al prezzo esorbitante di 20.000 miliardi. L'ENEL, a sua volta, negli ultimi anni, ha rivenduto all'egiziano Sawiris il pacchetto comprensivo della rete più i clienti, recuperando in parte i 20.000 miliardi sborsati alcuni anni prima. In conclusione,

Perché questo sintetico racconto, signor Presidente? In questo decreto, rappresentato come il decreto delle liberalizzazioni con Bersani difensore degli utenti‑consumatori contro i gruppi monopolistici che gestiscono la telefonia nel nostro Paese, c'è una norma contenuta all'articolo 1-*bis* in cui si dice che il Governo, per il tramite di un'iniziativa del Ministro delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può prorogare di 15 anni le autorizzazioni in capo alle reti delle telecomunicazioni. Questo vuol dire che due Ministri, al di fuori della trasparenza in questo caso necessitata nei confronti del Parlamento, possono autorizzare la proroga di 15 anni per i gestori delle telecomunicazioni (immagino la telefonia),

Egli dice: «non ho nostalgia per le vecchie concessioni affidate 20 anni fa, ma i rimedi tardivi spesso rischiano di produrre danni ancora maggiori». L'idea affascinante di far le gare di fronte a concessionari scelti con trattativa privata è un'idea che non vi porterà da nessuna parte perché non riuscirete a fare le gare entro l'anno. L'Unione Europea ha deciso che ai Paesi che non saranno in regola con il finanziamento e con l'intesa sul territorio

conclusione, signor Presidente, il ministro Bersani non ha contestato la mia precedente affermazione: la Genova-Milano non è né della FIAT, né dell'ENEl, ma di un consorzio di privati al cui capitale partecipano le banche. Sono già stati spesi 500 miliardi di vecchie lire. Mi dispiace

del decreto, recante misure urgenti a tutela dei consumatori, la promozione delle attività economiche e la conseguente nascita di nuove imprese, voglio in primo luogo sottolineare che si tratta di una provvedimento in continuità con altre misure approvate dal Parlamento nei mesi scorsi, in particolare con la legge n. 248 dell'agosto scorso - il cosiddetto Bersani-Visco - dove si affermò una nuova attenzione allo sviluppo economico, stimolando la concorrenza per allargare la base produttiva, intendendo le liberalizzazioni (questo è il punto che vorrei evidenziare) prevalentemente come strumento per facilitare l'acceso dei giovani al mercato, come salvaguardia dei diritti dei cittadini e come creazione di un nuovo rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, a partire dai Comuni e dagli enti territoriali. Ciò avviene soprattutto nel campo autorizzativo di attività economiche perseguendo il fine di una pubblica amministrazione che passa da un controllo burocratico di tipo quantitativo (distanze, parametri, limiti di accesso e aspetti cui faceva riferimento poc'anzi il ministro Bersani) ad uno qualitativo, basato sulla bontà dei progetti e sull'interesse pubblico. Questo è

ha determinato - come dimostrano i dati relativi - che la nascita di nuove attività di commercio e di somministrazione hanno contribuito grandemente alla riqualificazione dei centri urbani. Ieri i taxi, i panificatori e l'abolizione delle commissioni; oggi le ricariche telefoniche, i parrucchieri, i barbieri - per adeguarsi anche ai nuovi orari richiesti dalle esigenze delle donne e degli uomini nelle città che cambiano - le guide turistiche, le autoscuole, eccetera. Insomma, la semplificazione della nascita delle imprese è un tema affrontato oggi in questo decreto in termini di comunicazione unica al registro delle imprese

di nuovi impianti produttivi, assumendo - ecco il tema centrale - al posto dei controlli burocratici due grandi priorità strategiche per lo sviluppo economico ed occupazionale: in primo luogo, la valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle sue vocazioni, dei suoi beni culturali e dei suoi prodotti; in secondo luogo, l'occupazione stabile a tempo indeterminato dei giovani, intesa come risorsa. Ecco perché la modificazione normativa degli istituti tecnici ‑ su cui si soffermerà più tardi, per il nostro Gruppo, la senatrice Cappelli è urgente ed importante - infatti è stata integrata nei contenuti del decreto - per superare la gerarchizzazione imposta dalla riforma Moratti, poiché afferma pari dignità fra le diverse tipologie scolastiche. È ben strano che la destra, da una parte, si lamenti che ciò sia poco e, dall'altra, sia tanto preoccupata di difendere privilegi o corporazioni. Parliamo, a tal riguardo, di altri aspetti importantissimi del provvedimento, già illustrati nel dibattito (come l'abolizione del costo di ricarica telefonica, la trasparenza delle tariffe aeree

Ho trovato, a tal riguardo, assai singolare l'argomentazione utilizzata stamane dal collega Ferrara di Forza Italia, il quale si preoccupa del mancato incasso IVA di due miliardi

fra affidamento *in* *house* a soggetti interamente pubblici e quello ai privati. Sia chiaro che tali misure da sole non bastano; tuttavia, sono importanti e tipiche di un Paese moderno, che guarda al futuro perseguendo l'innovazione e che vede il lavoro dei giovani come una risorsa per facilitare l'accesso.

con politiche strutturali di sviluppo, innalzando le pensioni minime, tutelando i ceti deboli e creando un sostegno ai redditi più bassi per contrastare la povertà. Quindi, è davvero urgente convertire il

il poco tempo a disposizione con parsimonia e con il dovuto rispetto per quest'Aula che vede partecipare a questo dibattito numerosi senatrici e senatori, tutti interessati a proporre, all'interno di questa discussione, il punto di vista proprio e degli elettori e dei cittadini che rappresentano, ai quali va detta - secondo noi - una grande verità, che questo non è un decreto per le liberalizzazioni. Questo è un decreto che muove alcuni timidi e piccoli passi su un percorso che dovrebbe affrontare, innanzitutto, le vere liberalizzazioni che servono a questo Paese che riguardano i grandi servizi pubblici, le grandi rete strategiche, che riguardano tanto altro e diverso dal fatto che forse potremmo beneficiare di leggere con maggiore dovizia d'informazione i prezzi della benzina o che dovremmo rallegrarci del fatto che i parrucchieri e le parrucchiere potranno aprire i loro saloni anche di lunedì senza più rispettare le tabelle che un tempo avevano l'obbligo di rispettare. Ho ascoltato con attenzione, in particolare l'accalorato intervento del ministro Bersani che ha voluto richiamare alcuni princìpi - alcuni di questi condivisibili sul tema delle liberalizzazioni alle quali noi certo non ci sottraiamo, ma che sappiamo essere vere e utili alla democrazia proprio nella misura in cui riescono davvero a far ottenere a quei cittadini/utenti ai quali pensiamo quando parliamo di liberalizzazioni dei benefici reali. Ebbene, a partire dall'articolo 1 di questo decreto-legge - che riguarda le famose ricariche telefoniche che rischiano di diventare solo una forma di propaganda e di comunicazione che deve coprire quanto invece in questo decreto c'è che non va sia un lungo esempio di microliberalizzazioni e di presunte liberalizzazioni che non serviranno al nostro Paese. Gli utenti delle grandi reti di telefonia mobile scopriranno presto che nulla sarà cambiato nella loro bolletta perché le reti telefoniche sostituiranno al piccolo maltolto, o ben tolto, delle tessere prepagate l'aumento delle tariffe. Quindi, Quindi, per noi nulla cambierà. Come non cambierà quasi niente nel sistema economico del nostro Paese se le parrucchiere potranno restare aperte di lunedì. Potremo parlare davvero di liberalizzazioni, invece, quando affronteremo i temi veri delle liberalizzazioni che sono quelli che citavo prima, prima, quelli che a noi interessano e sui quali troverete il consenso del centro-destra. Su queste operazioni di comunicazione e propaganda non potrete mai ottenere il nostro appoggio e il nostro voto di fiducia vedrà, ancora una volta, dire no a iniziative di questo Governo che, come la storia dimostra anche in questi giorni, non vengono condivise dai due rami del Parlamento: sono iniziative di un Governo che tira diritto per la sua strada, che spesso entra a gamba tesa in alcune situazioni e in alcuni settori - molti di questi economici - arrecando grandi danni, e che poco si preoccupa del futuro economico di questo Paese che passa, certo, anche attraverso il processo di liberalizzazioni, che non vuol dire privatizzazioni. Ma per realizzare le liberalizzazioni bisogna porre al centro di queste gli unici davvero interessati, cioè gli utenti.

Noi, quando abbiamo varato la riforma Moratti, eravamo partiti da alcune considerazioni importanti. Innanzitutto, dalla considerazione che l'istruzione tecnica è fondamentale per il nostro sistema produttivo produttivo e, tuttavia, gli istituti tecnici da vent'anni a questa parte perdono iscrizioni. Perdono iscrizioni perché sono carenti nei contenuti, nei programmi, non si sono adeguati alle importanti trasformazioni tecnologiche

nostra riforma é che l'accesso all'università deve presupporre una preparazione culturale solida, non può avvenire per chiunque a prescindere dal percorso pregresso, altrimenti si creano illusioni che poi vengono amaramente frustrate.

alla legislazione precedente, perché l'obbligo scolastico si può adempiere anche nella formazione professionale regionale, in quelle scuole che danno semplicemente una qualifica. Allora dove sta la differenza? Solo nel

l'istruzione tecnica venga rafforzata. Intanto, non vi sono risorse: la riforma deve avvenire a costo zero. Francamente, prendere atto che una maggioranza che nella passata legislatura chiedeva addirittura investimenti di 8 miliardi di euro per il finanziamento della scuola superiore,

in contraddizione, peraltro, con emendamenti presentati alla Camera. E allora, o il Governo chiarirà con un prossimo provvedimento questo passaggio, oppure rischiamo un indebolimento dell'istruzione tecnica, che viene in qualche modo assimilata all'istruzione professionale. una istruzione professionale che presuppone due anni di istruzione generale, dopodiché, negli altri tre anni, ci saranno formazione professionalizzante, laboratoriale,

un peggioramento del nostro sistema di istruzione superiore. Certo, probabilmente una riforma siffatta ha anche deluso le aspettative di quella sinistra radicale che voleva la cancellazione *tout court* della legge Moratti: abbiamo visto come molti aspetti della riforma Moratti rimangano, abbiamo visto come addirittura sull'obbligo scolastico vi sia la stessa, identica fotografia della situazione preesistente con, tuttavia, alcune confusioni che andrebbero chiarite quantomeno in sede interpretativa. Dovevate rifare la scuola italiana, dovevate guardare

in verità, nel tempo a disposizione avrei voluto richiamare l'attenzione del ministro Bersani su alcune contraddizioni che ho rilevato nel provvedimento in esame

prima doveva essere il secondo decreto sulle liberalizzazioni, poi si è parlato di modernizzazioni; in realtà, il buon Bersani si è fatto scippare molta parte e si è fatto inserire nel maxiemendamento - lo hanno già detto molti colleghi prima di me una pseudoriforma della precedente riforma Moratti, nonché altre norme, dalla revoca delle concessioni a tante altre ancora,

quali risalgono al 1860, e questo non ci fa onore come parlamentari, perché vuol dire che legiferiamo troppo e male. Vorrei mettere in evidenza all'ottimo ministro Chiti che in questo provvedimento si vanno a toccare centinaia di norme di provvedimenti diversi e questo è un fatto gravissimo, che rende sempre più difficile in Italia l'applicazione corretta delle leggi.

Presidente, direi che in senso teatrale stiamo assistendo ad una commedia, scritta dal presidente Prodi, in cui gli attori sono i vari Ministri;

i quali si assumono anche loro alcune responsabilità, in qualche modo consentendo che questa commedia abbia troppe rappresentazioni, come quella odierna, abbastanza scadente ed offensiva per le vere prerogative dei parlamentari, che sono quelle di intervenire con proposte di modifica. A noi senatori oggi ciò non è consentito. Abbiamo assistito in Commissione industria ad una sceneggiata, abbiamo fatto finta di iniziare l'esame degli emendamenti, peraltro equamente presentati: metà dalla maggioranza e metà dall'opposizione. Vi rammento che anche per la stessa legge finanziaria, in quest'Aula, il numero degli emendamenti cosiddetta maggioranza di centro‑sinistra era praticamente uguale a quello degli emendamenti presentati dal centro-destra. Allora, devo pensare che avete una ancor più forte opposizione interna rispetto a quella visibile attraverso gli organi di informazione

intervengo soprattutto per esprimere il disagio, credo non solo mio ma di tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione, perché in questo ramo del Parlamento, un provvedimento così complesso e articolato non è stato esaminato. Abbiamo avuto in Commissione industria pochissime ore Lo dico con molta franchezza: non è serio per le istituzioni democratiche del nostro Paese. Ci rimettiamo tutti. Allora, ho voluto capire di più sul perché siamo arrivati ad avere questa situazione incresciosa per le istituzioni, le nostre istituzioni. ho sentito oggi pomeriggio il ministro Bersani - bravissimo, abilissimo - dare disponibilità al confronto, al dialogo e alla collaborazione su temi importanti come quello delle liberalizzazioni.

tempi. Qualche minuto fa, ho sentito un collega di Rifondazione Comunista dire: per noi «liberalizzazione» significa «semplificazione». allora ho capito il perché della strozzatura di questo dibattito. Vorrei dire al collega di Rifondazione Comunista che liberalizzare significa dare più spazio, più libertà economica alle imprese private in un libero mercato: significa la parola liberalizzazione. La semplificazione è una cosa diversa. Allora, mi è sorto il dubbio, credo legittimo, che si sia voluto strozzare questo dibattito perché probabilmente proprio qui al Senato si temeva un problema nella stessa maggioranza, visto un così palese disaccordo sul concetto fondamentale di cosa significa liberalizzare. Significa dare più spazio alle libertà economiche private in un libero mercato:

Un Paese democratico ha diritto a un libero dibattito, soprattutto su temi così importanti; non possiamo approvarli nel giro di poche ore senza alcun confronto. Per quanto

scuso per la brevità e per l'esempio irriverente: perché i ladri vanno a rubare quando è notte? Per non farsi vedere.

alla TAV, abbiamo ascoltato tante motivazioni. Di fatto, con questo intervento si mortifica uno Stato di diritto;

se occorreva una legge ordinaria per parlare di informazioni. Sarebbe stato sufficiente un semplice regolamento per semplificare la vita degli italiani e delle industrie che devono poi far fronte a tali disposizioni.

in Parlamento, ma soprattutto gli italiani, siano d'accordo sulle vere liberalizzazioni, ossia dare più spazio e libertà a chi opera nel mercato. Ho sentito ancora il collega di Rifondazione: i problemi li abbiamo sulle grosse, le vere liberalizzazioni, come i servizi pubblici locali, le poste, le ferrovie, le energie, la liberalizzazione dai vincoli burocratici enormi che esistono nel nostro Paese, del mercato e della competizione nel campo dell'università, una forma di liberalizzazione. Queste sono le vere liberalizzazioni che daranno davvero una spinta alla competitività. Sostenere che con i barbieri e con i facchini si possa migliorare la competitività del nostro Paese mi sembra un'affermazione un po' azzardata; quindi, e mi dispiace che non sia sia presente il ministro Bersani, potrei dire che piuttosto che una lenzuolata di liberi servizi, di liberalizzazioni, al massimo si tratta di un pannolino.

le liberalizzazioni sono una strada obbligata per il futuro del nostro Paese, in un mondo sempre più interdipendente. Potremmo dire che liberalizzazione è oggi il nuovo nome della competitività nel campo economico e nel campo della vita sociale. Scopo di un Governo che intenda farsi carico dei problemi sociali del suo Paese è quello di avviare con decisione questo percorso di liberalizzazione, essendo attento a regolare il quadro complessivo del mercato, che non può essere un mercato senza regole: libero non significa senza regole, ma ben ordinato e capace di tener conto delle diverse esigenze che si sovrappongono e interagiscono tra loro nel quadro di una società composita e complessa come quella italiana, ed europea più in generale, del nostro tempo. La ripresa della domanda interna viene incontro alle attese dei consumatori, e cioè di tutti noi, in qualche modo, e delle nostre famiglie; la ripresa della capacità d'impresa attraverso la concorrenza viene incontro all'esigenza dell'economia globale, che ha sempre più bisogno che i vari Paesi, le diverse economie, tanto più quelle più avanzate e industrializzate, interagiscano e si confrontino tra loro, dicevo prima, in un quadro ordinato anche a livello sovranazionale. Non si può negare che la volontà del Governo Prodi, sin dai suoi primi atti nella tarda primavera dello scorso anno, sia stata in questa direzione e con questa determinazione. Si tratta di aperture troppo timide, si tratta di argomenti che dovevano essere affrontati con più decisione e con più incisività? Siamo di fronte a semplici certificazioni amministrative, come si sente dire e abbiamo sentito dire anche adesso dai banchi dell'opposizione? Quand'anche fosse vero, collega Stanca e colleghi dell'opposizione, il vostro argomento proverebbe troppo, come si dice, perché è del tutto evidente che liberalizzare, nel nostro Paese, dove stratificamente si sono succedute corporazioni a corporazioni e protezioni a protezioni, significa anzi tutto ridurre, anche partendo da situazioni modeste, i lacci e lacciuoli della burocrazia, quelli che pesano di più, anche dal punto di vista percettivo, della percezione che se ne ha, nei confronti delle esigenze delle famiglie, delle singole persone, dei singoli lavoratori, dei singoli produttori. C'è stato un ruolo positivo delle corporazioni in tempi lontani, c'è stato un ruolo positivo di una protezione industriale ed economica in tempi di svalutazioni facili e di competizioni più accentuate e diverse da quelle attuali, ma oggi i tempi sono diversi, e qui è l'invito che dai nostri banchi viene al Governo a procedere con lena sulla strada positivamente imboccata dai provvedimenti del ministro Bersani e dei suoi colleghi - che, essendo io un parlamentare un po' all'antica e quindi girando sul territorio che mi ha eletto (spero lo facciano tutti i colleghi), ho incontrato, in queste ultime settimane,

È giusto, è bene che emerga questa domanda dai cittadini, è bene che chi pensa di essere colpito nella sua posizione di attività professionale, commerciale o quant'altro colpito nel senso di essere costretto a modificare le proprie abitudini - dai provvedimenti di liberalizzazione, non reagisca rifiutando il confronto e l'accettazione di quanto oggi disposto, ma chieda che quanto disposto nei confronti della sua categoria sia esteso il più rapidamente possibile alle altre. È questo il dovere che abbiamo, ma allora è evidente che i provvedimenti anche parziali del ministro Bersani e del Governo sono destinati ad innescare - e mi auguro che ciò avvenga il più rapidamente possibile - un circolo virtuoso, perché determinano l'attesa di ulteriori provvedimenti e quindi di meccanismi in grado di svecchiare la nostra economia, di svecchiare i rapporti sociali e commerciali all'interno del nostro Paese e di farci presentare più pronti alle sfide dei prossimi anni e decenni, che sono poi le sfide dell'innovazione e a fare meglio e sempre di più. Non ci si può fermare di fronte all'avanzare del progresso e delle nuove esigenze, né si possono rallentare, con una visione miope, da cicale che difendono il proprio recinto, senza comprendere che le generazioni future avranno comunque altri recinti più ampi di fronte a loro. Ricordo sempre che nella mia Regione, la Liguria, un tempo Sanremo e la Riviera dei fiori non erano territori in cui si coltivavano fiori; vi si coltivavano limoni, utili alla Repubblica di Genova per combattere lo scorbuto sulle sue navi.

Ciò spinse gli abitanti di Sanremo ad abbandonare le coltivazioni dei limoni e a scegliere un altro tipo di coltivazione, quella dei fiori, una scelta che ha fatto la storia del Novecento di quel territorio. allora che non bisogna mai avere l'atteggiamento di chi ha paura dell'innovazione e del nuovo. Certo, occorre contrattare, occorre concertare la possibilità di regole che garantiscano la sopravvivenza di coloro che sono inseriti in determinati circuiti di carattere produttivo, economico e sociale, ma occorre andare andare avanti con decisione su questa strada. Il Governo lo sta facendo e il nostro invito al Governo è di continuare con lena su tale percorso. Al riguardo, per concludere, richiamo l'attenzione del signor Ministro sull'ordine del giorno che porta la mia firma e che concerne due delle categorie interessate

da ogni parte d'Europa e del mondo. Da questo punto di vista, l'ordine del giorno chiede al Governo di proseguire sulla strada della liberalizzazione del settore in questione e, nello stesso tempo, di avviare tavoli di concertazione affinché l'intero settore, anche dal punto di vista della tutela dei lavoratori e di coloro che, spesso sottopagati, sono impiegati in tale veste, sia garantito nel modo migliore e più adeguato. In questo senso, confermo che esprimeremo la convinta fiducia al Governo su tale provvedimento. PRESIDENTE. Signor Presidente, senatrici e senatori, giunge al voto finale questo disegno di legge, che la propaganda mediatica definisce pacchetto delle liberalizzazioni e che questa opposizione, in forte *deficit* di argomentazioni, tenta di immiserire. come dice lo stesso titolo del provvedimento, si tratta di misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza e lo sviluppo dell'attività economica. Un provvedimento che avvia la nascita di un nuovo Paese - un Paese di cittadini, non di sudditi - e che raggruppa una serie di provvedimenti, piccoli ma significativi, per le persone che vivono una vita normale e che in questo momento è appesantita da difficoltà e da incomprensibili regole e costi. Tra questi provvedimenti ve ne è uno, quello che si compendia nell'articolo 13, che concerne l'istruzione pubblica, che ha caratteristiche particolari; in realtà, esso è difficilmente riconducibile alla *ratio* degli altri, per argomento, contesto e anche per la densità delle questioni culturali, politiche e ordinamentali che sottende. Si tratta di una norma che interviene strutturalmente, e spero definitivamente, sul sistema dell'istruzione e che assume una rilevanza che non è stata assolutamente colta nel dibattito parlamentare, anche se alla Camera, con il lavoro in Commissione e tramite emendamenti, si è intervenuti ad ampie mani sulla materia, migliorando il testo iniziale. Il provvedimento è, quindi, necessario e urgente. Restituisce il maltolto, restituisce al sistema nazionale della pubblica istruzione e alla gestione nazionale del Ministero l'istruzione tecnica e professionale, cancellando quella parte della riforma Moratti che la collocava nel secondo canale della formazione superiore, quello della formazione professionale con gestione regionale. Un canale di serie B, cui destinare i figli e le figlie delle classi popolari, in un'idea di società in cui il sapere alto, quello critico e complesso, è destinato a chi se lo può permettere, perché è merce e non è bene comune, non è diritto universale. A chi non può rimane le scuola finalizzata al lavoro, quella dell'abilità, del fare, della manualità, che magari prepara ad un lavoro precario. La riforma Moratti, insomma, metteva fine all'onda lunga del Sessantotto nella scuola, quando nelle centocinquanta ore i metalmeccanici non volevano solamente ottenere il diploma di licenza media, ma volevano anche accedere ad un sapere non immediatamente spendibile nel lavoro, come la musica e la filosofia. Noi, con l'articolo 13, riapriamo questa partita e questa speranza, in un contesto difficile e più complesso, anche perché l'obiettivo è meno esplicito e più forti e potenti gli avversari. In questo articolo vi è l'idea del rilancio dell'istruzione tecnica e professionale come punto forte della società e della conoscenza. Da un lato, vi è il riconoscimento della funzione storica che questo settore ha avuto, non soltanto nell'economia italiana e nel suo sviluppo, ma anche nella storia della cultura italiana, nell'estensione del diritto allo studio, nell'innovazione didattica e pedagogica, nella ricerca di un nuovo modo di fare scuola che produca nei giovani di oggi passione ed interesse, nella creazione di una nuova intellettualità diffusa e di massa. Dall'altro lato, vi è l'idea della possibilità di superare oggi in modo definitivo, a partire dall'occasione storica dell'innalzamento dell'obbligo a sedici anni e della definizione del biennio unitario; di superare il dualismo gentiliano fra le due culture, quella umanistica e quella tecnica e scientifica,

e che su questo si misuri oggi la politica lo si capisce anche dal fatto che gli anticipatori e i sostenitori della Moratti sfidano la Costituzione e il Governo, rilanciando il suo progetto senza mediazioni, come sta facendo in Lombardia Formigoni. Per questo diciamo che l'articolo 13 del decreto è positivo, necessario, ma assolutamente insufficiente e anche ambivalente nella formulazione del rapporto tra istruzione professionale e formazione, sulla titolarità delle funzioni e sui compiti, sull'obbligo scolastico come diritto-dovere. Sappiamo che l'ambiguità riflette diversità di approcci anche all'interno dell'Unione, che possono essere risolti solo mettendo al primo posto gli obiettivi del programma dell'Unione e l'interlocuzione continua e attenta con le scuole, strada disattesa - a mio parere - a partire dalla finanziaria ad oggi. Alla fine, critichiamo quella parte dell'articolo 13 che autorizza e norma le erogazioni liberali. Pensiamo che le scuole si finanzino attraverso la fiscalità generale e che di tutto avevamo bisogno fuorché di questa innovazione.

Signor Presidente, pensavo di avere meno tempo a disposizione, ma, comunque, gli argomenti non mancano.

sono tanti, ma cercherò di non sprecarli. Il ministro Chiti è persona simpatica e gradevole e lo ringrazio della sua presenza in Aula, mentre mi rammarico del fatto che non sia presente il ministro Bersani. Prima, interrompendo il Ministro, ma senza

della liberalizzazione della vendita dei farmaci o della presunta liberalizzazione dei taxi - e di questo parleremo - c'è stata la ciccia vera della stangata fiscale del ministro Visco in apertura di legislatura.

Quanto poi alla potenziale liberalizzazione dei mercati prevista nel provvedimento, Presidente, devo ricorrere ad una citazione: *Timeo Danaos et dona ferentes*, diceva Laocoonte ai Troiani, quando i Greci regalarono il cavallo di Troia attraverso cui espugnarono la città.

che, a suo giudizio, il mercato non avrebbe offerto una potenziale concorrenza sull'abolizione del costo di ricarica, spingendo in tal modo il Governo

Tutti coloro che hanno un po' di dimestichezza con la telefonia mobile ricorderanno che alcuni anni fa un operatore, Wind, entrò sul mercato proponendo proprio quello che il Governo ha imposto oggi per legge,

quell'operatore con quella mossa non ha però ottenuto il successo che voleva conseguire, perché i consumatori, nella loro libertà di scelta, hanno preferito altri operatori che pure gravavano la loro tariffa del costo di ricarica.

il mercato è libero e sono i consumatori con i loro comportamenti oggettivi a determinare se un elemento che costituisce il prezzo è vessatorio.

per raccontare una bugia ai consumatori e dire, invece, la verità in Parlamento. Infatti, ieri in Commissione il sottosegretario Lettieri ha giustificato il fatto che la norma sull'abolizione dei costi di ricarica non richiede copertura.

ragione non c'è bisogno di copertura per il mancato introito di IVA e per la riduzione delle imposte sul reddito delle società che vengono a percepire 2 miliardi di euro di meno, non poco. meno, non poco. Eppure, il Governo ci ha risposto che non c'è bisogno di coprire questa presunta diminuzione di IVA e d'imposta sul reddito semplicemente perché la riduzione degli introiti dei gestori non ci sarà perché essi rimoduleranno le tariffe. Allora, è bene dire questo agli italiani e non prenderli in giro, ministro Chiti, dicendo che si è intervenuti a loro beneficio. Non si è fatto altro che un intervento a piedi uniti

si troverà a pagare di più rispetto a quando esistevano i costi di ricarica, proprio in virtù di questa rimodulazione dei prezzi forzosa e voluta dal Governo, che non sa e non vuole sapere come operano i mercati e come la loro libertà e la contrattualità

al di fuori e contro la legge. In questo caso si interviene con la stessa logica: si blocca per legge un elemento di composizione del prezzo, non sapendo che gli altri andranno liberamente e i consumatori da questo riceverebbero danni. Siete degli apprendisti stregoni; non mettete le mani sul mercato, perché non lo conoscete! Avete familiarità con i Gosplan, con le programmazioni, ma con la libertà di mercato, con l'impresa, con la contrattualità che c'è tra consumatori e imprese non ci sapete fare. Non conoscete neanche come andava; non sapete neanche che un gestore ha offerto le sue ricariche senza costi e il mercato le ha rifiutate. Avete toccato con lo scorso provvedimento i tassisti dicendo che, grazie alla vostre misure, sarebbe aumentato il numero dei taxi disponibili, non avremmo avuto problemi nelle ore di punta e avremmo finalmente consentito l'apertura della professione di tassista ai giovani. Il risultato è quello che abbiamo tutti sotto gli occhi a Fiumicino. All'aeroporto di Fiumicino oggi c'è il caos totale nel settore dei taxi, perché non è aumentato di una macchina, le tariffe sono totalmente amministrate e se si prende un taxi proveniente da Roma si pagano 40 euro, mentre se lo si prende proveniente da Fiumicino se ne pagano 60, in base agli accordi che i Comuni hanno stipulato

usando la benzina come prodotto civetta e, quindi, non ricaricandovi utili per attrarre consumatori, offrirebbe dieci centesimi in meno al litro.

alle attese. Abbassate le tasse, se volete che i consumatori, i cittadini, gli operai e i pensionati, stiano meglio. Gli avete tolto la *no tax area* e pensate di ricompensarli abolendo i 5 euro di ricarica che poi diventeranno 10 euro, quando utilizzeranno il cellulare? Questa è pura propaganda demagogica. La realtà dei fatti, signor Ministro, signor Presidente, è che avete un disegno strategico di controllo dell'economia italiana e state dando a tutti un segnale

che aveva, quello di intervenire sui criteri di formazione dei prezzi. Fissate i prezzi per legge e che cosa fate in questo provvedimento? Quello che vi interessava: la controriforma della scuola, che nulla ha a che fare con la liberalizzazione (perché semmai era quella riforma che liberava risorse e energie per la scuola), e la revoca delle concessioni TAV, perché tra i concessionari non ci sono i vostri amici e non siete riusciti a piazzarli neanche tra i subappaltanti, le cooperative di costruzione non hanno avuto spazio. Forse mirate a quello: se riuscirete a indire alcune gare (cosa di cui dubito, perché la vostra maggioranza è contro lo sviluppo delle infrastrutture del Paese, come lo è stata nei cinque anni del nostro Governo)

la nostra partecipazione agli atti legislativi e la nostra passione nell'attività e nella vita politica vengono mortificati e messi a dura prova di pazienza.

mi pare che non siano da sottolineare come ostruzionismo, ma come effettivo lavoro e costruzione di un qualcosa (di regole, di leggi, di normative)

di fiducia vi risolve il problema dei tempi e del tempo, ma non fa un bel servizio al Parlamento - soprattutto al Senato - né al Paese ed ai cittadini. a cosa ci porta a questo documento, com'è già stato sottolineato anche da altri colleghi? La sensazione è che siate dei novelli Robin Hood, solo

oltretutto si ritroveranno in busta paga decine, anzi, centinaia di euro in meno, nel corso del prossimo anno, per effetto della vostra legge finanziaria. Liberalizzate certe categorie (i barbieri, le parrucchiere, i facchini e via dicendo), ma non toccate i grandi monopoli di Stato, i grandi servizi, le esclusive

radiografate persino i conto correnti bancari, non solo dell'azienda ma anche della famiglia, dei titolari. Introducete l'etichettatura dei prodotti, ma permettete che si smaltiscano le scorte senza definire tempi e metodi, chissà cosa succederà. Siete abituati a fare i duri con i deboli e i fragili con i forti, lo avete fatto nei giorni scorsi con i militari in Afghanistan. I nostri militari li trattate

interrompete le relazioni con le Regioni, abbandonate la formazione professionale al suo destino,

Il Ministro diceva in questi giorni che era stufo di vedere la scuola italiana continuamente nel tritacarne e che i fatti che emergono dalle cronache riguardano una piccolissima parte di studenti e di insegnanti. È vero, ne sono convinto. Ma nel tritacarne la sta mettendo lui. La riforma La riforma della scuola l'ha fatta in finanziaria ricevendo 20 deleghe specifiche che potrà usare come vuole! Una parte della riforma della scuola è stata inserita in questo decreto-legge di liberalizzazione. Cosa c'entra?

Li abbandonate, non ne tenete conto. Né accettate il principio fondamentale che anche attraverso il lavoro si può arrivare alla cittadinanza attiva,

quello che dovreste o vorreste essere. signor Ministro, onorevoli colleghi, anche questa legge di conversione del decreto-legge del 31 gennaio scorso viene imposta agli italiani con un voto di fiducia. Il ministro Chiti si è dichiarato amareggiato, ma noi siamo più amareggiati di lui per l'ulteriore richiesta di fiducia. Ieri, la delegazione UDC ha rappresentato al Presidente della Repubblica, tra le altre cose, questo abuso dei decreti-legge *omnibus* e il ricorso alla fiducia, soprattutto al Senato, per il frequente decorso dei 60 giorni alla Camera. Di fatto, si sta introducendo in modo surrettizio un sistema monocamerale, quello della Camera, constatando la ricorrente blindatura dei decreti. L'UDC nei prossimi giorni denuncerà *con* forza questo punto. Detto questo, signor Presidente, affrontiamo quella che è una «legge manifesto» per il centro-sinistra. Essa è l'ennesima legge truffa, che passa con il marchio contraffatto delle liberalizzazioni, ma, gratta gratta, si trova un altro pezzo di riforma della scuola e poi la revoca delle concessioni rilasciate dalle Ferrovie dello Stato alla società TAV S.p.A. per la realizzazione dell'Alta velocità.

e di questa materia c'è poco, se non alcuni adempimenti imposti dall'Unione Europea e poi della tutela dei consumatori, che ripropone correzioni di norme del precedente decreto Bersani e attua sollecitazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. È una "lenzuolata" a strisce, è un decreto *omnibus* che cerca di recuperare consenso elettorale, non ha alcuna incidenza sul sistema economico nazionale, non incide di un decimale sul PIL; non crea posti di lavoro, perché con razionale cannibalismo sociale, quelli che crea li compensa poi con quelli che cancella; aumenta l'offerta dei servizi a danno degli *standard* di qualità; invade le competenze regionali e locali che reagiranno con forza come già preannunciato; mortifica ancora una volta il Parlamento con due voti di fiducia, il settimo alla Camera, nonostante la maggioranza abbia oltre 60 parlamentari in più dell'opposizione, e l'ottavo al Senato. Complessivamente 15. Auspichiamo che il diciasettesimo vi porti sfortuna. fiducia perché vi è stato l'ostruzionismo dell'opposizione: non è vero per l'UDC, per espressa affermazione soprattutto della vostra Marina Sereni, ma non è vero nemmeno per il resto dell'opposizione, perché lo stesso ministro Chiti poc'anzi ha ricordato che su 35 modifiche ben 21 erano sottoscritte dall'opposizione e questo vuol dire che c'è stato un apporto costruttivo da parte

Se questo decreto-legge è importante, non potete mortificare così il Parlamento, ed il Senato in particolare. Se mortificazione non c'è, perché non è importante, allora abbassate i toni trionfalistici usati anche dal ministro Bersani poco fa. Non è vero che fa risparmiare le famiglie italiane, non è vero che rompe antiche incrostazioni che penalizzano il Paese e la sua economia, non è vero che stimolano le imprese a crescere, non è vero che si investe sul capitale umano e tecnologico del Paese. Di liberalizzazioni - c'è scritto - si tratta solo per "alcune" attività economiche, com'è scritto nella *rubrica legis* dell'articolo 10; la prima è quella di acconciatore e di estetista, ossia di quelli che alcuni ancora chiamiamo «barbiere» e «parrucchiere», che vedono rimossi i limiti della distanza minima e del numero chiuso e non hanno più l'obbligo della chiusura del lunedì. La seconda è quella di pulizia, disinfezione e facchinaggio: chiunque adesso può svolgere detta attività, aprendo così una guerra tra poveri, soprattutto extracomunitari. La terza è quella della guida turistica e dell'accompagnatore turistico, dove non occorre più alcuna autorizzazione preventiva, soprattutto da parte delle Regioni, aprendo così un contenzioso con le stesse Regioni, come dicevo, già preannunciato. La quarta è quella relativa alla gestione delle autoscuole, dove non occorrerà più il limite della popolazione e dell'estensione territoriale, che garantivano gli *standard* di qualità delle prestazioni. La quinta è l'abolizione dell'albo italiano dei consulenti del lavoro, stante la procedura d'infrazione contro l'Italia avviata dalla Commissione europea. Qui finiscono le liberalizzazioni. Nella «lenzuolata » di Bersani ci sono, però, i cosiddetti risparmi per le famiglie. Vediamoli. Ricariche telefoniche: divieto di applicare contributi aggiuntivi nonché prevedere limiti temporali delle carte prepagate. Grande truffa mediatica. Infatti quel 90 per cento di italiani che usa carte prepagate si troveranno compensati sulle tariffe telefoniche il contributo fisso anticipato. Lo ha riconosciuto, questo, in Commissione, lo stesso sottosegretario Lettieri alla Camera. Al gestore di telefonia mobile sarà assicurata la stessa entrata e al consumatore la stessa spesa: dove è il risparmio? L'unica soddisfazione sarà una maggiore trasparenza. Non è un risultato da far alzare la voce. I mutui sulla prima casa: divieto di clausole penali per estinzione anticipata e portabilità del mutuo. Non mi sembra, anche qui, il caso di alzare la voce. Anche qui sarebbe stato interessante se aveste applicato la norma ai contratti di mutui in corso, ma non si è potuto fare e qui si scopre il trucco. Infatti, già molte banche non applicano la penalità per l'estinzione anticipata del mutuo, a condizione però di qualche decimale di maggiorazione del tasso d'interesse, quindi ai tassi praticati non si potevano fare sconti sui presunti costi di estinzione anticipata. Quello che prima era facoltativo e valutava liberamente il cittadino che contraeva il mutuo, adesso diventa obbligatorio con le banche. Un bel regalo alle banche, le quali si rifaranno sui maggiori tassi d'interesse a danno dello stesso cittadino che a questo punto non può più scegliere come poteva fare prima. Anche qui, quale risparmio per le famiglie e i cittadini? Si è parlato di trasparenza di prezzi e tutela del consumatore.Vediamo anche qui che cosa propone la «lenzuolata» di Bersani. Primo *spot*: informazioni adeguate, anche in forma comparata, circa i prezzi del carburante praticati sulle tratte autostradali e sulle strade di primaria importanza, ponendole a carico del gestore della rete autostradale e stradale. È una dichiarazione di principio. Si tratta di vedere con quali strumenti si attuerà e la capacità di accesso che avranno gli automobilisti. Anche qui, nessun richiamo contro la pubblicità ingannevole. Secondo *spot*, tariffe aeree: divieto di fare offerte e messaggi pubblicitari di tariffe arbitrariamente scomposte tra il costo di vettoriamento e costi aggiuntivi che danno luogo a pubblicità ingannevole. Terzo *spot*: indicazione chiara, leggibile e indelebile della data di scadenza dei prodotti alimentari, soprattutto quelli deperibili; tale obbligo c'era già, si rende solo più esplicito: anche qui, occorre alzare la voce? Piuttosto, come va interpretata la norma per i prodotti in commercio a lunga conservazione alla data di scadenza dei 180 giorni della vecchia normativa? Chi pagherà i danni dei magazzini pieni di prodotti ancora validi? Altro che risparmio e trasparenza, qui si fa propaganda politica - *spot*, appunto - sulle spalle di chi lavora! Altro aspetto: concorrenza e tutela del consumatore nei servizi assicurativi. Qui ho l'impressione che il centro-sinistra se la suoni e se la canti. Infatti si modifica una norma che ha introdotto il ministro Bersani con il decreto-legge n. 223 del luglio scorso. È chiaro l'errore fatto l'estate scorsa, quando si limitò il divieto di distribuzione esclusiva solo alle polizze RC auto. Adesso si rimedia estendendo tale divieto anche alle polizze relative a tutti i rami danni. Meglio tardi che mai. Ma anche questo ditelo sottovoce, perché noi ve lo avevamo già detto, e anche a voce alta, l'estate scorsa. Un altro *spot* di questo decreto-legge è quello della nascita di un'impresa in solo giorno. Avete rubato all'onorevole Capezzone un'iniziativa che aveva una qualche consistenza politica, perché razionalizzava una serie di procedure e autorizzazioni per impiantare un'attività imprenditoriale. Il peso della burocrazia voi invece lo spostate da prima a dopo, ma non lo eliminate o riducete. Il peso dei controlli inutili e delle vessazioni amministrative lo invertite: invece che svilupparlo prima, lo sviluppate dopo l'apertura dell'attività, ma rimane tutto intero. È il gioco delle tre carte per guadagnare un po' di pubblicità tra chi non sa. Se un'impresa nasce iscrivendola in un giorno nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, costringendola a fare comunque tutte le successive pratiche inutili, rimane per voi il problema di far vivere poi questa impresa. Con la pressione fiscale e lo *stress* da adempimenti burocratici successivi, la condanna a morte è tra le cose possibili. Non parlo della rottamazione perché pure voi del centro-sinistra vi vergognate a parlarne, trattandosi di una correzione dei commi 224 e 225 dell'articolo 1 della finanziaria per il 2007, che vi ha visti troppo sbilanciati verso le aziende automobilistiche, in modo grave ed incomprensibile. Al di là del titolo di questo decreto‑legge, il vero peso specifico, sul piano politico, è rappresentato dalla controriforma sulla scuola e dalla revoca delle concessioni alla TAV spa. Con la cancellazione dei licei economici e tecnologici della riforma Moratti e il ripristino degli istituti tecnici e professionali, fate fare un passo indietro alla riforma e per di più con un decreto-legge su cui metterete due fiducie. Lo dico soprattutto a chi ha criticato la riforma Moratti, fatta senza l'assenso dell'allora opposizione, come si è detto. Se la riforma della scuola non andava fatta con l'autosufficienza dell'allora maggioranza della Casa delle Libertà, nemmeno la controriforma però va fatta pezzo dopo pezzo, con decreti ministeriali e decreti‑legge imposti con il voto di fiducia. Su questa linea ci sono pezzi dell'attuale maggioranza che la pensano come noi: penso ai socialisti e agli stessi comunisti italiani. La scuola italiana è in difficoltà e voi inserite confusione a confusione. La vostra faciloneria nelle decisioni è pari all'irresponsabilità dei comportamenti. Altra norma irresponsabile in questo decreto è quella dell'articolo 13, di revoca delle concessioni TAV spa, soprattutto per le tratte Milano-Verona, Verona-Padova e la linea Milano-Genova, di cui ho parlato questa mattina in sede di pregiudiziale di costituzionalità. Le concessioni furono date quando Romano Prodi era Presidente dell'IRI e furono revocate già nel 2000 dal centro-sinistra e riconfermate nel 2002 con il cosiddetto collegato alle infrastrutture da parte del centro-destra. L'idea della riconferma delle concessioni alla TAV si fonda sulla circostanza che lo stesso ente Ferrovie dello Stato, partecipando a società che progettano e realizzano linee ed infrastrutture ad alta velocità, con lo sfruttamento economico delle stesse infrastrutture, recuperi il capitale investito dalla stessa società. In sostanza si opera come per anni ha operato la società Autostrade quando era pubblica. La soluzione scelta dal centro‑sinistra, invece, fa saltare tutto il sistema con l'aggiunta dell'aggravamento finanziario dovuto all'indennizzo per risarcimento danni derivante da fatto lecito: appunto, la revoca. Quindi non solo il sistema imprenditoriale italiano sarà probabilmente escluso dai lavori, ma sarà anche penalizzato dai danni che subirà per la risoluzione dei contratti *ope legis.* Nemmeno impegnandosi si riuscirebbe a fare tanti danni su più fronti, così come avete fatto con questo decreto. La nostra fortuna è che la vostra produzione legislativa è minima e i danni sono limitati; diversamente ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli. Avremmo voluto dare una mano sulle liberalizzazioni, ma quelle vere, quelle sui servizi pubblici locali. Le contraddizioni e le liti dentro la maggioranza ce lo impediscono e il disegno di legge è ancora fermo in Commissione. Volevamo recuperare i contenuti in questo decreto, ma, di fatto, ci è stato impedito alla Camera e ci è impedito al Senato con la blindatura del provvedimento. I costi di luce, acqua, gas, trasporti pubblici, smaltimento e raccolta dei rifiuti sono le tariffe che pesano sui cittadini, senza alcun riscontro sul rapporto qualità-prezzo e senza concorrenza, perché gestiti dai monopoli locali delle ex aziende municipalizzate. Tali tariffe colpiscono tutti indistintamente, soprattutto pensionati, operai e disoccupati, che non possono fare a meno dei servizi pubblici essenziali, ma riformarli colpirebbe di più le clientele e il vostro sottogoverno nell'80 per cento degli enti locali che amministrate. tali riforme non le farete mai e vi limiterete a leggi manifesto e *spot* pubblicitari, che servono ad avere qualche respiro elettorale, ma non all'Italia e ai suoi cittadini. Perciò, il nostro è un no chiaro e ragionato; non è un no pregiudiziale. La vera sfida che impone una seria apertura dei mercati riguarda la separazione delle reti (tutte le reti) dalla gestione dei servizi; la separazione della rete da Telecom Italia e la liberalizzazione delle frequenze UMTS, rimuovendo, soprattutto, i vincoli urbanistici che permettono la salvaguardia dello *statu quo ante* a favore della stessa Telecom Italia; l'abolizione del CIP6 e la revisione del sistema dei certificati verdi; la privatizzazione del BancoPosta; la privatizzazione di Trenitalia e la separazione della rete ferroviaria; realizzazione dei gassificatori, il riconoscimento delle associazioni professionali e il restringimento delle materie riservate agli ordini professionali, rivedendone la legislazione. L'UDC vi sfida su queste vere liberalizzazioni di sistema. Con la legge Biagi abbiamo liberalizzato il mercato del lavoro rispetto alle timidezze del cosiddetto pacchetto Treu, e il 6,4 per cento dell'attuale livello di disoccupazione ne dimostra la bontà. Abbiamo regolato il mercato del risparmio dopo gli scandali Cirio e Parmalat con la legge sul risparmio e ce la vengono a copiare dall'estero. Potremmo proseguire con la riforma della scuola, delle procedure sul fallimento, delle procedure del codice civile e della previdenza. Togliete Prodi, superate l'autosufficienza elettorale; aprite il Parlamento a nuove esperienze di Governo; abbiate il coraggio di superare questo bipolarismo inchiodato dai ricatti della sinistra massimalista; apritevi a maggioranze più ampie e facciamo le riforme che servono all'Italia. Uscite dal guscio e dalla logica di parte; fate gli interessi dell'Italia e non delle vostre piccole convenienze. Abbiate coraggio! Se rimetterete l'Italia al centro della politica, l'UDC la troverete. Questa è la nostra sfida. Diversamente, la nostra opposizione è chiara, netta, decisa, come su questo decreto. Presidente, sarò molto rapido. Avrei voluto confrontare le mie osservazioni con le tesi esposte dal Ministro

quella che revoca alla società TAV le concessioni per la progettazione e la realizzazione delle linee ad alta velocità non ancora cantierizzate, e precisamente quelle relative alle tratte Milano-Verona-Padova e Milano-Genova. Gli effetti di tali revoche, recita ancora l'ex articolo 12, si estendono a tutti i rapporti convenzionali stipulati da TAV spa con i *general contractor* che verranno liquidati previo accertamento e indennizzo delle spese realmente sostenute e «adeguatamente documentate». Ci sembra questo un provvedimento importante, volto a rendere maggiormente trasparenti le modalità di affidamento delle concessioni e che sembra comporterà comunque un risparmio rispetto alla previsione di spesa che il completamento delle opere, così come sono state immaginate, implicherebbe. Inoltre, sempre nell'ex articolo 12 vengono apportate modifiche alla legge n. 241 del 1990, stabilendo che la revoca di un atto amministrativo deve tener conto dell'esistenza e della permanenza di un interesse pubblico: un segnale di trasparenza importante, secondo noi, un primo passo per iniziare a ricostruire una relazione di fiducia tra i cittadini e chi li governa, per superare il sospetto, e in verità spesso più che un sospetto, che quelle grandi opere su cui si è fondata una parte consistente della politica del precedente Governo, più che nell'interesse pubblico fossero realizzate e favore di gruppi di interessi lobbistici. Ci auguriamo che tale provvedimento rappresenti un'assunzione di responsabilità, che il Governo si impegnerà, d'ora in avanti, a verificare le reali disponibilità finanziarie, i preventivi economici e gestionali per ogni singola tratta e l'applicazione effettiva delle norme in materia di valutazione degli impatti ambientali, affinché venga definitivamente superato quel «modello TAV» fondato su false previsioni, sottostima di costi, sovrastima di ricavi, finanziamenti privati inesistenti, fantasiose opere, spesso irrealizzabili, e che ha comportato invece la nota crisi nelle casse delle Ferrovie e fatto accumulare 13 miliardi di euro di debiti a carico del bilancio dello Stato. Certo andrebbe, secondo noi, riaperta la discussione per rivedere l'intero progetto Alta velocità e Alta capacità, poiché i dati emersi anche nelle audizioni dei vertici delle Ferrovie dello Stato, che abbiamo audito in 8a Commissione, ci dimostrano come i costi di queste linee siano, in Italia, molto elevati: 32 milioni di euro per chilometro, contro i 10 milioni della Francia, e quelle in progettazione e realizzazione addirittura 45 milioni di euro contro i 13 della Francia. Ci chiediamo se ne valga la pena, a fronte dei gravi disagi che tanti cittadini, lavoratori pendolari, studenti, sono costretti a sopportare a causa delle precarie condizioni in cui versa la rete ferroviaria ordinaria. Ecco, secondo noi questo decreto-legge è il primo passo verso il riavvicinamento tra la politica e i bisogni concreti delle persone, ma sarebbe necessario andare oltre, invertire la rotta e ricostruire una relazione vera con i territori, con quei cittadini che continuano a rivendicare a gran voce un ruolo da protagonisti, che chiedono trasparenza e aderenza ai bisogni reali, con quei cittadini che, proprio come nel movimento «No TAV», sono capaci di immaginare un futuro diverso, migliore per tutti,

Signor Presidente, nei miei pochi minuti non ripeterò le cose che i miei colleghi hanno già detto, ma toccherò solo alcuni passaggi, soprattutto in relazione all'intervento del ministro Bersani di oggi Anch'io voglio sottolineare, intanto, il fatto che queste così sbandierate liberalizzazioni in realtà riguardano settori assai marginali dell'economia del Paese, e soprattutto non daranno minimamente quel ritorno, in termini di risparmio per le famiglie, così come detto invece dalla maggioranza, dal Governo e dal Ministro. A proposito delle ricariche telefoniche non aggiungo altro a quanto detto semplicemente, per ammissione dal Governo stesso, non ci sarà nessuna diminuzione di costi, quindi l'argomento si chiude già da sé. Per quanto riguarda le assicurazioni, ricordo che questo decreto va a colpire solo gli agenti assicurativi, quelli sul territorio, con una serie di adempimenti in più che in realtà porteranno pochissimi risparmi alle famiglie, ammesso che ne possano portare, perché comunque ormai il margine di tali lavoratori è veramente ridotto da anni all'osso e caricare di ulteriori adempimenti burocratici questi uffici porterà semplicemente alla chiusura di molti di loro senza incidere minimamente sul prezzo e sul costo delle tariffe, quanto riguarda le assicurazioni intese come compagnie assicurative, di fatto, in questo decreto non c'è assolutamente nulla. Per non parlare poi dei benzinai. Questa è una norma veramente

Quand'anche i benzinai lavorassero gratis, per le famiglie ci sarebbe un risparmio di non più di 15-30 vecchie lire al litro, quando lo Stato guadagna 1.700 lire di tasse per ogni litro di benzina e con l'aumento del petrolio degli ultimi anni ha ha incrementato i propri introiti, perché non ha almeno avuto il buonsenso, come abbiamo indicato sia nella scorsa che in questa legislatura, di fare una tassazione al litro e non una tassazione al costo per litro, che perlomeno avrebbe mantenuto su livelli accettabili i prezzi dei carburanti. Per quanto riguarda poi i barbieri, se con questa norma mettiamo a posto il Paese ne siamo contenti, vorrei però anche qui sottolineare con un po' più di serietà la contraddizione in termini. Qui c'è una maggioranza che ha gran parte dei suoi voti poggiati sulla sinistra e sulla sinistra radicale antagonista, quella che lotta da anni per le 35 ore, se non meno, per i lavoratori. Con le grandi *holding* dei parrucchieri, che evidentemente non ci sono, ma il piccolo barbiere di paese, se non vuole chiudere perché magari la coop del paese vicino ha messo un negozio di parrucchiere al suo interno con parrucchieri da essa dipendenti, a tenere aperto il suo negozio sette giorni su sette per non perdere i clienti. clienti. State veramente dividendo il Paese tra i superprotetti dalla vostra ideologia e quelli che, sempre secondo la vostra ideologia, devono scomparire, perché sono uomini liberi,

con questo provvedimento e anche con quelli dell'anno scorso, sempre del ministro Bersani, di cui andiamo a parlare adesso. Sulla scuola e la TAV non aggiungo altro a quanto già detto, voglio solo sottolineare che veramente non so se definire più ridicolo o offensivo che al Parlamento italiano si porti una riforma della scuola con un decreto‑legge sulle liberalizzazioni che al Senato staziona solo 48 ore. Credo che non sia serio, soprattutto da parte di una maggioranza di sinistra come la vostra, che della scuola, dell'istruzione e della cultura giustamente ha fatto da sempre una propria bandiera. Sulla TAV aggiungo poche considerazioni a quanto già detto, solo per sottolineare un attimo le questioni importanti. Voi di fatto bloccate, come noi avevamo molto facilmente preventivato in campagna elettorale, ogni opera pubblica importante, oltre a compiere un atto assolutamente illegittimo. Non so come potete pensare di bloccare i contratti in corso, come potete pensare di andare ad affrontare i contenziosi, le penali, gli anni di tribunale che questa vostra scelta andrà a comportare; oltre al discorso non trascurabile, visto che siete sempre una maggioranza di sinistra, che in questo giorni il sindacato sta protestando contro il Governo per il blocco dei cantieri, che solo tra Lombardia, Piemonte e Veneto

Lo stesso per le farmacie. Adesso vendiamo la cibalgina alla coop, così tra un po' avremo anche in Italia le statistiche degli iperconsumatori di farmaci inutili. Non si è preso neanche

Gli anglosassoni - gli americani, per intenderci - quando fa comodo sono il demonio internazionale e, sempre quando fa comodo, diventano riferimento per le liberalizzazioni. per le liberalizzazioni. È stato, invece, veramente offensivo quando ha detto che il cittadino non deve essere un suddito. Ricordo al ministro Bersani che io non mi sento meno suddito perché dalla prossima settimana potrò andare dal barbiere anche il lunedì pomeriggio,

Signor Presidente, mi soffermerò semplicemente su un tema di questo decreto: la revoca delle concessioni della TAV. Ho ascoltato prima la collega Palermo, che probabilmente o era disattenta quando l'amministratore delegato e il presidente delle Ferrovie sono intervenuti in Commissione qualche giorno fa, o ha detto una mezza verità.

non ci sono i soldi. La capacità di questo Governo è quella di tassare gli italiani e di non avere i soldi per realizzare grandi opere pubbliche.

che tutto questo fa piacere ai Verdi e a Rifondazione Comunista, in particolare, perché non si realizzeranno più opere pubbliche in Italia. Siamo passati da un Governo del fare ad un Governo del non fare, che oggi è diventato Governo del disfare. Credo che il primo punto che bisogna lasciare agli atti sia che per i danni che verranno richiesti e saranno pagati dallo Stato italiano ci debba essere una responsabilità personale dei Ministri che hanno portato avanti e sottoscritto le revoche di queste concessioni. Vorrei citarne una: mentre alcune tratte, due in particolare (la Milano-Verona e la Verona-Padova), sono ancora in fase di strutturazione del progetto,

ma messo in atto lo sciopero, perché 9.000 lavoratori del settore - ma è evidente che questo vi interessa poco - hanno già perso la possibilità di cassa integrazione e altri 6.000 rischiano nei prossimi mesi di perdere il posto di lavoro. 15.000 lavoratori: non vi interessa. Forse vi interessa di più la cosiddetta mobilità lunga per la FIAT, la classe padrona, che da sempre è abituata a socializzazione le perdite, cioè assegnarle a carico dallo Stato, ed essere molto libera sugli utili, cioè incassarli.

Signor Presidente, Ministro, colleghi, il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, al nostro esame fa parte del pacchetto di misure sulle liberalizzazioni con il quale il Governo intende provvedere all'eliminazione di svariate barriere normative all'accesso al mercato del lavoro, che colpiscono in particolare i giovani; all'introduzione di maggiore concorrenza nel mercato economico interno; ad una maggiore tutela del cittadino consumatore. Di questo pacchetto, lo ricordo, oltre al decreto-legge che stiamo trattando fa parte anche il disegno di legge delega sul completamento della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, per il risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, con alcune parti, originariamente in esso contenute, entrate in vigore con l'ultima legge finanziaria. Vi sono, poi, il disegno di legge delega per il riordino dei servizi pubblici locali, al centro di un approfondito dibattito in Commissione affari costituzionali; il disegno di legge delega in materia di professioni intellettuali; il disegno di legge sul riassetto dell'Autorità indipendente di regolazione, vigilanza e garanzia dei mercati; e, infine, il disegno di legge relativo alle misure di agevolazione delle attività produttive e commerciali e a misura per il cittadino consumatore. Un'organica serie di provvedimenti legislativi di fronte ai quali il centro-destra si è esercitato in un ampio spettro di rilievi critici, di vario spessore politico. Da parte di alcuni esponenti del centro-destra, anche qui al Senato, si è arrivati a parlare di demagogia, di populismo, di norme farraginose e fuorvianti, in un crescendo che ha raggiunto toni derisori, financo offensivi. In tutto questo fuoco di sbarramento, due critiche meritano una risposta, pur nella limitatezza dei tempi. La prima riguarda i tempi ristretti per l'esame del decreto qui in Senato: siamo d'accordo. Il fatto è però che i tempi ristretti a disposizione del Senato sono conseguenza diretta di quanto avvenuto in sede di esame del decreto alla Camera dei deputati. Mi riferisco evidentemente alla scelta dell'opposizione di ricorrere all'ostruzionismo, una scelta non motivata né motivabile con l'argomento di chiusure della maggioranza e del Governo. Tant'é che quando sono state avanzate proposte ed osservazioni, quando cioè l'opposizione ha voluto e potuto scendere sul terreno del confronto parlamentare, il decreto è stato emendato, come del resto è stato riconosciuto nel corso del dibattito alla Camera sia da esponenti dell'opposizione sia dallo stesso Ministro qui in Senato. Certo, se al posto del confronto si sceglie la strada dell'irrisione e dell'ironia (come ha fatto, ad esempio, di par suo l'onorevole Tremonti il quale in verità, nella precedente legislatura, ha fatto ampio sfoggio di ironica creatività nella gestione della sua delega ministeriale) o addirittura si parla, come ha fatto questa mattina il senatore Ciccanti, di decreto «capolavoro di imbecillità politica», allora credo francamente che venga vanificata ogni possibilità e/o volontà di confronto costruttivo. Il voto di fiducia diventa, a questo punto, una scelta inevitabile per impedire la decadenza del decreto, con le conseguenti negative ripercussioni che si avrebbero.

o rendere più trasparenti taluni comportamenti, adottati dai gestori della telefonia mobile, Internet e televisione, dalle autostrade, dalle banche, dalle assicurazioni e dalle compagnie aeree, che comportino costi ingiustificati a carico dei consumatori e meritevoli di essere rimossi; era inevitabile che il risultato sarebbe stato quello di un pacchetto che attenesse a vari aspetti della legislazione vigente. Tuttavia non si può certo affermare, come purtroppo è stato detto, che siamo in presenza di norme farraginose. Il decreto-legge n. 7 del 2007 costituisce il punto di arrivo di un ampio processo politico-legislativo il cui asse strategico è la stimolazione della crescita economica, l'aumento dell'attività della concorrenza e l'abbattimento dei costi per le famiglie e le imprese. Questo provvedimento contiene misure che intervengono sull'efficienza del sistema Paese, eliminando e semplificando procedimenti amministrativi. La difesa del cittadino consumatore, un cittadino titolare di doveri, ma anche di diritti - come ha sottolineato il ministro Bersani nelle sue conclusioni - è l'altro punto fondamentale di questo processo di liberalizzazioni. un pacchetto di interventi che erano stati già previsti nel programma di Governo, sulla base del quale abbiamo chiesto il consenso dei cittadini per governare il Paese, e contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011. Del resto, l'unica norma realmente ultronea concerne, all'articolo 13, le nuove disposizioni per la scuola; proprio quelle norme su cui, come è del tutto evidente, si è maggiormente realizzata in qualche misura la convergenza tra maggioranza e minoranza. Il punto, signor Presidente, è comunque che questo rilievo (che si tratti cioè di un decreto *omnibus*) ci lascia molto perplessi. Posso capire, in questa come in altre occasioni, che vi sia una sorta di inevitabilità dell'opposizione di turno all'avanzamento di tale rilievo. L'abbiamo fatto anche noi; tuttavia, la perplessità resta tutta, perché è questo un rilievo critico che potremmo aspettarci da un cittadino arrivato nel nostro Paese per la prima volta in questi giorni, non certo da chi nella scorsa legislatura, in tutti i cinque anni della sua durata, ha fatto ricorso ripetutamente a decreti *omnibus* per le materie più disparate. Su questo si potrebbero fare innumerevoli esempi, voglio qui ricordare solo quanto è successo in un settore a me particolarmente caro, cioè quello della Protezione civile, dove, con l'inserimento di norme ultronee in vari provvedimenti, si è smantellata l'Agenzia; si è ripetutamente intervenuti sull'organizzazione del Dipartimento e sulle sue funzioni, sul suo ruolo, spesso in spregio ai richiami della Corte costituzionale e alla dichiarazione di infrazione avanzata dalla Commissione Europea. Viceversa, questo decreto contiene misure che nascono da da segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Credo di poter dire che sia la prima volta che un provvedimento del Governo nasce anche a seguito delle segnalazioni di singoli cittadini e di associazioni. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo sia molto facile fare dell'ironia sulla semplificazione delle procedure per l'inizio d'attività per acconciatore ed estetista (e comunque vicino al Senato da alcuni giorni è stato aperto un negozio grazie a queste norme). Reputo altresì che sia nel vero chi ha sottolineato come in questo decreto siano contenute norme di puro buon senso che in un Paese normale sarebbero state oggetto di normali provvedimenti amministrativi.

avanzate in settori a forte domanda ed aperti a grandi innovazioni tecnologiche e organizzative; norme volte a ridurre il costo dei servizi alle imprese ed ai lavoratori,

Liberalizzare è un concetto ed un impegno politico che è stato totalmente assente nell'agenda dei vari Governi Berlusconi. Esso è un concetto ed un impegno che era ben presente (come ho già detto) nel programma di Governo dell'Unione per la XV legislatura, come lo è stato nell'azione dei vari Governi di centro-sinistra alternatisi nella XIII legislatura, come lo sono oggi - e ne sono il filo rosso che li unisce in un tutt'uno organico - nel pacchetto Bersani. Allora, non sorprende se Jean-Philippe Cotis, capo economista dell'OCSE, osservatore molto critico in passato verso il nostro Paese, abbia dichiarato come riportato su «Il Sole 24 ORE» del 14 febbraio - che le riforme presentate dal Ministro Bersani sono «un punto cruciale per stimolare la concorrenza e quindi la crescita economica (...) un piano coraggioso e ambizioso che noi appoggiamo. Lo sforzo di liberalizzazione è di importanza capitale per l'Italia, da anni penalizzata da (...) costi troppo elevati nei servizi e costi domestici che sono negativi per la concorrenza». E poi, ancora: «Le liberalizzazioni sono molto importanti per ristabilire le competitività del *made in Italy* e stimolare la crescita interna».

Governo, colleghe e colleghi, anch'io vorrei intervenire sulla parte relativa alle norme sulle tratte ad alta velocità Milano-Genova, Milano-Verona e Verona-Padova. Le norme che il Governo propone sono una svolta - a mio giudizio e del Gruppo dei Verdi - importante, utile e positiva per fare ordine nella realizzazione delle infrastrutture ferroviarie che servono al nostro Paese, per aumentare il mercato e la concorrenza negli appalti pubblici, per ridurre i costi degli investimenti e, quindi, risparmiare risorse pubbliche (che, peraltro, non abbiamo o sono assai scarse), e per scegliere con criterio le infrastrutture effettivamente prioritarie. Certo, stiamo parlando di una vicenda assai lunga che ha origini nel 1990, quando si affidò senza gara l'intero sistema Alta velocità, a pochi giorni dall'entrata in vigore della direttiva che, dal 1° gennaio 1993, avrebbe obbligato tutti a effettuare le gare. Si disse allora (in parte si continua a sostenere) che si doveva proteggere il sistema delle imprese italiane, al quale era riservata la realizzazione dell'Alta velocità. Se questa motivazione probabilmente reggeva allora e aveva le sue buone ragioni, non regge più adesso, quando nel 2007 parliamo ancora degli stessi progetti, che non sono stati realizzati

Non credo che nel 2007 difendere il sistema delle imprese italiane significhi continuare a proteggere affidamenti senza gara effettuati nei primi anni

ormai in fase conclusiva, di cui abbiamo urgentemente bisogno); il fatto che la TAV, che era privata al 60 per cento, è diventata pubblica nel 1998, perché si è ammesso che nessun privato nessun privato è un ente di beneficenza e che per realizzare infrastrutture con siffatte caratteristiche servono ingenti risorse pubbliche (così come hanno fatto tutti i Paesi europei) e che sarà RFI dello sfruttamento economico. Infine, voglio ricordare che anche il progetto è cambiato ed è diventato dedicato non solo ai passeggeri, ma anche alle merci, e fortemente interconnesso con i nodi. Fu a seguito di questo lungo e difficile percorso - che, da un lato, avviò

vennero revocati i contratti delle tratte non iniziate, le stesse di cui stiamo parlando (la Milano-Genova, la Milano-Verona e la Milano-Padova). Ma cosa accade nel 2001, quando il centro‑destra vince le elezioni e va al Governo del Paese? Arriva il ministro Lunardi che, insieme alla legge obiettivo, propone - per far presto, tra le tante cose, con la legge n. 166 - anche la restituzione a trattativa privata, evitando, quindi, le gare, per le tre tratte di cui stiamo parlando.

finanziamento. Per questa ragione, sono assolutamente inaccettabili le grida del centro‑destra che anche in quest'Aula riecheggiano. Se quel postulato, infatti, si fosse rivelato autenticamente vero e realizzato, non staremmo qui a discutere della revoca, nel 2007, delle tre tratte: sono state revocate, infatti, ma il problema è che il modello proposto dal centro-destra non ha funzionato. Dobbiamo ammetterlo:

da un lato, tutti - soprattutto noi Verdi - dobbiamo compiere passi in avanti, anche il centro-destra dovrebbe ammettere che il suo modello non ha funzionato: semplificazioni eccessive, niente gare e risorse che poi non sono nemmeno state poste a protezione della realizzazione.

perché non erano state nemmeno rispettate le autorizzazioni ambientali prescritte. Questi, quindi, sono purtroppo gli unici cantieri aperti e chiusi molti anni fa. Pertanto, vorrei che svolgessimo un ragionamento serio:

Non c'è dubbio che la materia è di grande delicatezza: stiamo parlando di un rapporto tra Stato e soggetti privati. Vorrei però far presente che il provvedimento di revoca

stato impensabile tornare indietro perché il contenzioso sarebbe stato rovinoso per l'interesse pubblico e quindi per l'interesse del sistema Paese. In questo caso,

dunque, sono le risposte di merito che volevo dare a chi dice che stiamo azzerando unilateralmente dei contratti. Qui ci sono norme primarie, norme derivate, ci sono convenzioni e non atti integrativi, clausole di salvaguardia - naturalmente, ovviamente e giustamente - delle spese effettivamente

In tal senso difendo la norma contenuta all'interno del provvedimento sul quale il Governo chiede il voto di fiducia. Un altro argomento che viene utilizzato è che si perdono risorse europee pure sono state assicurate. Vorrei ricordare che Bruxelles non ha deciso assolutamente nulla in ordine ai finanziamenti e che proprio per le difficili situazioni della finanza pubblica europea

privilegiate le tratte transfrontaliere a cui sarà destinato fino al 30 per cento di contributo. Ripeto, siamo nel campo delle proposte e non della certezza. Per l'Italia si dice apertamente che le due tratte che hanno qualche *chance* di essere finanziate sono il valico del Brennero e il valico della Torino-Lione che, peraltro,

serissimo. A chi dice che perderemo soldi per la Milano-Genova, dunque, ricordo che siamo nel campo delle ipotesi. Non ci sono risorse assegnate, c'è una corsa incredibile al finanziamento europeo in cui, a mio giudizio, la Milano-Genova non è una infrastruttura che ha possibilità di essere finanziata. Certezze: nessuna.

Voglio solo citare il dato che si riferisce al tema delle gare (poi parleremo del resto nelle sedi opportune): le mancate gare - dicono le Ferrovie - pesano per l'incremento dei costi dal 14 al 20

Napoli-Bari, un progetto di cui abbiamo bisogno. Potremmo parlare anche, ad esempio, della tratta Padova-Mestre; adesso non ho il tempo di discutere del nodo di Bologna, che ho approfondito e in effetti presenta dei problemi, però tutti i casi dimostrano che là dove si espletano le gare i costi tendono ad abbassarsi.

corretto ed equo, in cui siano date reciproche e adeguate garanzie, ma proprio per questo riteniamo utili per l'interesse pubblico le norme presentate in materia di Alta velocità: per aumentare mercato e concorrenza,

mi conferma nel senso di avvilimento e frustrazione che, come parlamentare, provo nel non aver potuto affrontare un dibattito così importante per il nostro sistema Paese, essendo espropriato,

Ebbene, laddove sono state attive le concessioni, ad esempio a Genova e a Napoli, sono stati portati avanti i lavori di costruzione delle metropolitane; al contrario, a Roma, dove si è spenta la concessione e ci si è illusi di poter procedere attraverso appalti, il sistema è stato bloccato per dieci anni e si è ripartiti, con la linea B1, attraverso un sistema che assomiglia a quello delle concessioni, grazie all'appalto integrato introdotto proprio dalla legge n. 166, cui ha fatto riferimento la senatrice Donati. Per la linea C, si è comunque ritenuto di dover ricorrere al sistema del *general contractor.*

dati mancanti. A mio parere, se realmente non si volesse abbandonare - e non si voleva abbandonare - il sistema della trasversale dell'Alta velocità, andava ritrovata proprio all'interno dei contratti la possibilità di scioglimento per evitare che si innescassero (come accadrà) contenziosi inevitabili, non tanto e non soltanto dal punto di vista economico, ma dell'uso della proprietà intellettuale delle progettazioni, è questo il punto. La verità è che con questo provvedimento si è fatto il fatto il passo ulteriore di spegnimento della politica delle grandi opere; è come se noi avessimo una macchina per andare da Roma a Milano e avessimo messo sabbia nel carburante e, non avendo il coraggio di dire che non vogliamo andare a Milano, diciamo semplicemente che la macchina non cammina. Questo mette addirittura in ombra quello che è stato fatto con il DPEF l'anno scorso sulla Val di Susa dove, derubricando la Val di Susa dalla legge obiettivo e dovendo necessariamente, a questo punto, andare in via ordinaria sulla valutazione di impatto ambientale, non avremo più assolutamente i tempi per stare all'interno della *quick short list* europea e quindi dovremo rinunciare non soltanto ai finanziamenti europei, ma ai sistemi facilitativi per fare quel tipo di raccordo. È lo spegnimento del Corridoio 5, è lo spegnimento della politica dei corridoi, è la politica, come ha detto il senatore Martinat, del disfare, di cui oggi A me dispiace che questo avvenga senza avere la possibilità in quest'Aula di dibattere in modo serio ed approfondito di tali argomenti vitali e cruciali per il sistema Paese. Invito tutti su questo, caro Presidente, a leggere le dichiarazioni dei sindacati nel documento della triplice. Leggo dal documento Fillea CGIL, CISL e UIL: «Il sostanziale blocco dei lavori e la revoca dei contratti per le nuove tratte Genova-Milano e la parte di Milano verso Venezia non pregiudica soltanto il completamento del sistema Alta capacità, ma mette in discussione il piano finanziario che sosteneva, e quindi significa buttare a mare 29 miliardi di lavori già eseguiti. La decisione del Governo di revocare per decreto i contratti da molti anni assegnati, se ha il pregio di recuperare un vizio formale di origine in quanto questi lavori erano stati assegnati senza gare, non chiarisce le motivazioni del risparmio, poiché il contenzioso che si aprirà sarà superiore ai benefici. Inoltre, è grave che il Governo non abbia definito i tempi delle nuove assegnazioni». Questo non lo dico io, ho citato letteralmente il documento di Fillea CGIL, CISL e UIL.

che la votazione per l'elezione della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, già prevista per la seduta antimeridiana del prossimo mercoledì 4 aprile, abbia luogo in altra data. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. **Ordine del